del suo Presidente. Vorrei essere rassicurato sul fatto che ella non possa rinunziare alla sua tutela personale. Sino ad oggi sono stato rassicurato dal fatto

Se non è possibile, significa che egli dice delle bugie anche su cose minimali, non soltanto sulle tasse o sui problemi dello Stato. Se invece non dice bugie, ho una preoccupazione: che lei possa rinunziarvi. E di questo vorrei essere rassicurato. Potrebbe esserci un'altra soluzione

ha trattato la questione con grande superficialità. Probabilmente la mia umile persona non è stata abbastanza e sufficientemente capace di fare opera di sensibilizzazione su un problema forte e umano

intervengo per esprimere solidarietà all'Arma dei carabinieri e più specificamente a quei giovani dell'Arma che

preferirono immediatamente scendere in piazza per le giornate dell'orgoglio e del bacio. Oggi sappiamo dalla magistratura inquirente

quella grande opera che ha la città di Roma, il Colosseo, e che forse non merita perché di sera diviene un ricettacolo di sporcizia e anche di atti sessuali svolti in pubblico. Mi permetto di segnalare ai tre Ministri del Governo, che molto poco

idee. Come i giornali hanno riportato con grandissima evidenza, è accaduto un fatto grave nello Stato che ospita il Parlamento europeo che quindi ha anche un qualche dovere in più rispetto agli altri Stati sovrani, poiché è chiaro che l'ospite gode anche di guarentigie millenarie, non soltanto di quelle relative allo *status* di parlamentare. È accaduto che in Belgio,

che il Governo italiano non si accontenti soltanto di questo intervento, ma solleciti il Governo belga a dare una risposta esaustiva ed esauriente

ha facoltà. BONFRISCO *(FI)*. Signor Presidente, ruberò pochi minuti solo per aggiungermi alla vibrata protesta del senatore Barbato che ha segnalato all'Aula lo spiacevole incidente accaduto a Pola.

che la nostra rappresentanza in quel Paese forse dovrebbe essere più attenta nel garantire

che forse, se si dimenticasse di qualche sua simpatia titina e si ricordasse maggiormente che si tratta di cittadini italiani che hanno subito un'ingiustizia e una violenza gratuite,

all'estero, in un Paese che dovrebbe essere insieme con altri la culla della democrazia, è stato invece oggetto di un ingiustificato arresto. Vorrei che il ministro D'Alema, con la stessa rapidità

Onorevoli colleghi, ieri, 11 settembre, ricorreva il 6° anniversario degli attentati di New York e Washington. Ricordo che lo scorso anno cerimonia molto partecipata presso la Sala Zuccari per ricordare il 5° anniversario dell'accaduto. A nome dell'Assemblea del Senato e mio personale, ho inviato ieri all'ambasciatore degli Stati Uniti Ronald Spogli un messaggio per rinnovare in modo non formale la nostra amicizia e vicinanza al popolo americano insieme alla condanna per un evento tanto drammatico quanto inumano. Quel giorno, che ricordiamo bene anche per le immagini incredibili e strazianti trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, la follia assassina dei terroristi falciò in pochi istanti circa 3.000 vite innocenti. A tutti va oggi il nostro commosso ricordo e alle loro famiglie il nostro affettuoso pensiero. Vi prego di osservare un momento di raccoglimento.

ha confermato il calendario di questa settimana e ha approvato il nuovo calendario fino al 20 settembre 2007. La prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 18 settembre, saranno innanzitutto esaminati congiuntamente il decreto-legge sulla sicurezza stradale e il disegno di legge recante norme sulla stessa materia, con modalità che saranno definite dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Gli emendamenti sui due provvedimenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani. Riprenderà poi, sempre nel corso della prossima settimana, la discussione sul disegno di legge recante delega sugli enti di ricerca, avviata prima della sospensione estiva. Sulla base delle richieste avanzate oggi dai Gruppi, la Presidenza prenderà contatto con il Governo per organizzare un dibattito sulla revoca e sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della RAI. Gli ulteriori argomenti della prossima settimana e di quelle successive saranno definiti dalla Conferenza dei Capigruppo, nella prossima riunione, da convocare per martedì 18 settembre, alle ore 12.

la nostra Costituzione prevede espressamente: «Ogni cittadino italiano può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale». Questa è una delle libertà fondamentali che sono iscritte nel nostro dettato costituzionale. Un sistema di trasporti efficiente non significa soltanto libertà, rappresenta anche, in relazione alla sua qualità, un requisito essenziale per riconoscere la civiltà di una Nazione e il grado di sviluppo di un Paese. Coloro che sono addetti a tale tipo di servizio, tanto a livello pubblico quanto privato, devono avere - e sottolineo con forza questo "devono" - rispetto e perizia nel proprio lavoro, almeno quanto un medico deve averne per i propri pazienti. Ci sono ancora troppe conquiste da compiere, tappe da raggiungere, obiettivi da centrare nel nostro Paese per poterlo definire europeo a tutti gli effetti. Molti di questi obiettivi sono proprio nell'ambito dei trasporti. Non a caso vorrei far partire questa mia denuncia proprio dall'annosa e penosa situazione di tutti quegli uomini, donne e studenti che si trovano costretti

Come possiamo anche solo pensare, quindi, di poterci confrontare con i nostri cugini d'Oltralpe o con i latini spagnoli? problema è molto grande. Un medico, sapendo che il suo operato produce inevitabilmente conseguenze non solo per il suo paziente ma anche sulle persone che gli sono accanto, idealmente e formalmente presta un giuramento a manifestazione del profondo rispetto dovuto per l'uomo, per la persona e per il suo microcosmo, intendendo per questo tutto ciò che ognuno di noi ha intorno, e siamo milioni di persone e milioni di microcosmi. Così, simbolicamente, anche gli operatori dei trasporti dovrebbero prestare una sorta di giuramento, poiché sono in grado di incidere o recare danno, come fanno spesso, alla vita dei cittadini che usufruiscono del servizio da loro reso. La mia mozione verte su una vicenda specifica che coinvolge negli ultimi anni il trasporto aereo nel nostro Paese, ma vuole anche ricomprendere il problema, molto più generale, che concerne l'intero sistema dei trasporti in Italia. È infatti oggi del tutto evidente la profonda crisi che attraversa il settore aereo italiano e la compagnia nazionale, che soffre di antiche scelte sbagliate. Pensiamo anche solo all'acquisto di aerei inadeguati e poi abbandonati nuovi negli *hangar*, inutilizzati per anni. Per non parlare poi della firma di contratti clientelari, con stipendi più consoni a piloti della NASA, che hanno portato alla formazione di caste di privilegiati. Questa categoria, presente anche in molti altri settori del nostro trasporto, si oppone con fermezza a qualsiasi tentativo di cambiamento oramai necessario ed inevitabile, facendo pagare allo Stato ed a ogni singolo cittadino italiano l'onere della sua sopravvivenza a volte dannosa. Se oggi, qui, in quest'Aula, potessimo invitare tutti gli italiani, sono assolutamente certo che ognuno di loro potrebbe raccontare una personale vicenda che li ha coinvolti nell'utilizzo di un mezzo di trasporto, e sono altrettanto sicuro che non si tratterebbe di vicende con un risvolto positivo o lusinghiero per il nostro Paese. Ho già fatto in premessa l'esempio dei pendolari, ma posso anche portarne uno personale che coinvolge quello che dovrebbe essere un fiore all'occhiello delle nostre ferrovie, l'Excelsior, che copre la tratta Roma-Milano, con il costo di un biglietto da *Concorde*, ma che di fatto fornisce un trattamento da pensione a due stelle. Più e più volte sono infatti stato testimone ed attore di proteste che puntualmente si concludevano con la sentita preghiera, da parte degli stessi operatori che prestavano il servizio, di attivarmi, in veste di parlamentare, affinché si ponesse finalmente rimedio a tale stato dei fatti. Visto che idealmente vi ho condotto attraverso il racconto di un'esperienza personale - e me ne scuso - su questa tratta, scendete con me a Milano e tentiamo di prendere una coincidenza all'aeroporto di Malpensa o Linate. Immaginiamo di essere ancora in piena estate: non sarà ugualmente difficile immaginare come tale coincidenza possa saltare, come fatalmente accade. Sarà capitato a molti di voi, come a moltissimi comuni cittadini, di essere vittima della cronica disorganizzazione dei nostri aeroporti ma, soprattutto, dell'atteggiamento del personale che, ritenendo di difendere quelli che oramai sono palesi privilegi, ricorre a mezzi scorretti attraverso regolamenti invece volti a salvaguardare la sicurezza del passeggero, utilizzati come un mezzuccio per ottenere una attenzione indotta. Parlo, naturalmente, dell'oramai tristemente famoso «sciopero bianco», che si esplica attraverso non una normale astensione dal lavoro, regolamentata dalla legge proprio per tutelare anche il cittadino-consumatore e non solo quello lavoratore, ma di una applicazione pedissequa e ottusa dei regolamenti stessi. È ora di dismettere la maschera da buonisti, da difensori ciechi dei lavoratori e di vestire quella da guida vera del Paese, assumendocene le responsabilità. Se non la smettiamo di nasconderci dietro falsi pretesti e passivismo clientelare, finiremo con il dare ragione al pennivendolo di turno che ciarla di caste inutili per il Paese, ed io aggiungo, soprattutto inutili per chi ha scelto l'impegno civile della politica pensando di dare un contributo al progresso del proprio Paese. Oggi sono qui per denunciare una pratica perversa, che ha prodotto notevoli disagi a molti cittadini italiani e stranieri, dei quali mi faccio idealmente portavoce, vittime di voli cancellati inopinatamente all'ultimo minuto, magari ad imbarco già effettuato, causato dal venir meno improvviso di un numero minimo di personale di cabina - come si dice nel regolamento - richiesto che, attraverso la denuncia di falsi malori, consente al comandante di chiedere, *ope legis,* la cancellazione del volo stesso immantinente. Se la cancellazione del volo fosse seguita ad uno sciopero regolarmente preannunciato e svolto secondo le previsioni di legge, il cittadino si difenderebbe, sarebbe in grado di tutelarsi e di organizzare nel modo migliore la propria vita ed i propri interessi. Ma quando il personale di cabina, con premeditata lucidità, impedisce una partenza sa perfettamente cosa comporta la cancellazione improvvisa anche di un solo volo (ma sono decine); sa perfettamente ed approfitta del disagio causato alle vite, agli interessi, agli affetti coinvolti per richiamare maggiore attenzione sulle proprie rivendicazioni, molto spesso ingiuste. Pensiamo, ad esempio, all'avvocato che non potrà presenziare all'udienza lungamente attesa e che, quindi, con lo zampino della farraginosa macchina giudiziaria, dovrà attendere un anno più per poter avere una nuova udienza, con un inevitabile nocumento tanto per la sua professione quanto per la vita delle parti coinvolte. O, ancora, immaginiamo l'accordo tra importanti aziende che salta per il mancato appuntamento o, ancor più, nel quotidiano, l'impossibilità di un ricongiungimento familiare o del godimento di ferie tanto Pensiamo alle famose coincidenze di cui parlavamo prima: quanti stranieri hanno perso la coincidenza per l'Olanda o per la Germania, dovendo pagare nuovamente il biglietto, sì poi rimborsato,

Quanti esempi ancora potremmo portare, più di 350 ogni singola volta che un aereo non si alza in volo per un comportamento scorretto e inaspettato

difesi e sono tutelati dalla Costituzione, ma che noi non facciamo valere. Non posso non pensare che in altri Paesi a simili comportamenti sarebbero seguiti seri provvedimenti contro gli autori, i quali senz'altro sarebbero perseguiti. Negli aeroporti italiani, però, la *via crucis* del passeggero non si sostanzia, purtroppo, solo nella cancellazione improvvisa dei voli o nella pessima qualità del servizio infine reso o, ancora, nella lentezza del trasporto stesso, ma anche - e ricordiamo cosa è accaduto solo lo scorso mese - nel furto e nella perdita dei propri bagagli. Mi amareggia dover affermare che questa è una realtà soprattutto italiana, in particolare alla luce della mia esperienza di voli internazionali che come ogni parlamentare mi trovo alcune volte ad intraprendere. Proprio pochi giorni fa mi sono ritrovato a far parte di una delegazione in visita nella lontana Cina. Ho così potuto personalmente verificare come, pur essendo quello un Paese dai forti contrasti politici e sociali, il servizio di trasporto di cui ho usufruito sia stato impeccabile: grande puntualità, coincidenze perfette e consegna celere, immediata e sicura dei bagagli per tutti e sei i voli consecutivi, sia interni che esterni, su cui abbiamo viaggiato. Inutile dilungarmi nel raccontare poi del trasporto ferroviario cinese, che vanta punti di eccellenza nell'alta velocità, che viaggia a più di 400 chilometri orari e passa su ponti sospesi e sotto i letti dei fiumi, come accade per il tratto sotto il Canale della Manica. A questo proposito voglio citare

«La TAV» - ha continuato il Ministro - «è un'opera necessaria per il Paese perché bisogna far capire di che cosa stiamo parlando: stiamo parlando di strutture ferroviarie necessarie». «Quando mi occupo della Val di Susa vedo» - ha detto il Ministro - «cittadini giustamente preoccupati a cui bisogna dare delle risposte e le stiamo dando». Secondo il Ministro, però, a quelle manifestazioni intervengono persone che poco c'entrano con il problema: «Vedo che partecipano i *no global* dei cosiddetti disoccupati organizzati di Napoli, i *no global* di Berlino, il movimento Arcigay di non so dove, e allora il vecchio Di Pietro direbbe: ma che c'azzecca tutto questo con la Val di Susa?». E ha ragione Di Pietro. La maggioranza prenda atto che non è in grado di risolvere questi problemi, che pure il Paese ha. E non dimentichi la maggioranza

di Messina. Cosa dobbiamo poter vantare oggi? Il lungo tratto su rotaia unica che collega o, per meglio dire, isola il Sud dal Nord? O l'abbandono delle azioni messe in campo dal precedente Governo, a cominciare dalla TAV? è assolutamente necessario che il Governo si impegni non solamente sul fronte degli investimenti (sicuramente indispensabili) e sulla rapida realizzazione delle opere strutturali fondamentali per portare il nostro Paese a poter competere con gli altri Paesi europei, anche solo per poter restare in Europa, ma anche a dettare norme cogenti e una disciplina quadro che riguardi il comportamento verso i terzi - come chiedo nella mozione sottoscritta da diversi colleghi difesa dei cittadini consumatori, che non sono oggetti, ma rappresentanti di una realtà personale e famigliare (il microcosmo al quale ho fatto riferimento) che le azioni

È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà.

tocca uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi: la crisi e il futuro dell'Alitalia. È in atto ormai da mesi la riflessione tra partiti, sindacati e associazioni che, proprio in questi ultimi giorni, si è concentrata sull'approvazione delle linee-guida

nella quale le parti hanno concordato sul trasferimento di 14 dei 17 voli intercontinentali da Malpensa a Fiumicino. La decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che l'*hub* di Malpensa non è di destinazione, ma di transito. Nel corso dei colloqui, inoltre, è stato chiarito che le ore di volo complessive non diminuiranno poiché ci sarebbe un aumento dell'impiego dei velivoli, e questo aspetto è stato apprezzato molto dai piloti che hanno espresso soddisfazione sulle decisioni assunte dal nuovo presidente Prato. alla luce di quanto appena descritto, la fase di emergenza scioperi che nei mesi scorsi ha fatto registrare nel settore del trasporto aereo fortissimi disagi per i viaggiatori, caos infernale negli aeroporti sia nazionali che internazionali, nonché ingenti perdite anche a livello economico, che si stima siano di molte decine di milioni di di euro, dovrebbe a questo punto rientrare. È d'obbligo ancora una breve riflessione: la questione della privatizzazione dell'Alitalia è ancora aperta. Notizie varie si susseguono anche in queste ultime ore: un'agenzia ha battuto la smentita dell'esistenza di «contatti in corso e ad altissimo livello» con Air France. Ad ogni modo, non è questa la sede più opportuna per entrare nel merito di una vicenda complessa per la quale il Governo e la società stanno lavorando con serietà alla costruzione di un progetto che salvaguardi il futuro della compagnia di bandiera, recuperando gli errori di gestione del passato. La riorganizzazione di Alitalia deve passare attraverso la ricerca di *partner* che puntino ad un serio risanamento dei conti e degli sprechi e su alleanze coerenti che sviluppino l'iniziativa industriale.

Signor Presidente, come Lega Nord Padania desideriamo sostenere l'iniziativa del collega Cutrufo e di altri

gradi. Il sistema di trasporti fa inevitabilmente acqua da tutte le parti. Vi è una grossissima difficoltà a mettere sul mercato un'azienda di Stato che a tutti i cittadini pesa enormemente. Non esiste un'impresa come Alitalia in questo Paese che realizza 2 milioni di euro al giorno di perdite: una fabbrica di debiti. Nel momento in cui si stabilisce che i cittadini italiani non possono continuare a pagare 2 milioni di euro al giorno per sanare il *deficit* di Alitalia, credo sia interesse di tutta la comunità trovare la formula giusta per far finire questa emorragia. Sembrava che alcune compagnie fossero interessate a subentrare

di un grosso piano di ristrutturazione aziendale. Questo vuol dire probabilmente che, a giudizio di qualsiasi imprenditore dei trasporti, vi è un problema di esuberi. Vogliamo Vogliamo salvare Alitalia in quanto tale o vogliamo salvare fino all'ultima pedina di Alitalia? Questo è il nocciolo del problema.

macchina Alitalia, ha fatto desistere il potenziale acquirente, che il giorno dopo ha ringraziato, ha lasciato il tavolo della trattativa e tutto ristagna come prima.

però dobbiamo anche evidenziare che questa macchina è disomogenea e disarticolata. Fatto 100 il volume di passeggeri che annualmente transita su Fiumicino,

La mozione, specificatamente, dice che non è possibile consentire ogni altro giorno che questi scioperi continuino a deteriorare la compagnia, a farla perdere, a renderla a renderla meno appetibile ad eventuali, nuovi, possibili o potenziali acquirenti e, a maggior ragione, che continuino a creare danni e disagi ai cittadini.

anche questi italiani, che non possono continuamente mettere mano alle tasche, perché nei costi complessivi dello Stato italiano c'è questo bubbone che, una volta

altri senatori e vorremmo anche rincarare la dose, richiamando alla massima responsabilità il sindacato, che non ha il solo e precipuo compito di tutelare i dipendenti Alitalia, ma tutti i dipendenti che pagano i debiti che Alitalia produce in questo Paese.

cominciare credo che sulla questione, come inevitabile, si stiano addensando tutte le problematiche che hanno travagliato e continuano a travagliare non tanto il sistema dei trasporti in Italia,

che, se applicate correttamente, portano obiettivamente alla cancellazione di molti voli e comunque a ritardarne tanti altri. Il punto di vista del Governo - raccogliendo con ciò lo spirito e anche la sostanza della mozione

Il Governo non sopravvaluta né sottovaluta quanto accaduto e condivide pienamente le preoccupazioni espresse nella mozione,

al Parlamento, al Senato in questo caso, o in sede di Commissione o in sede di Aula, come si riterrà opportuno procedere. C'è un'istruttoria in corso in merito alla questione della regolarità dei voli che cerca di distinguere quanto dipende da fattori tecnici, quindi non strumentali, da quanto dipende dalla volontà dell'uomo e, all'interno di questa, quali e quante organizzazioni sindacali - nell'eventualità che sia accertata una soggettiva responsabilità nel provocare tali ritardi o cancellazioni - appartengano a questa o quella sigla sindacale. Sono stati ravvisati parecchi punti di criticità sui quali forniremo una relazione compiuta. Per finire, vorrei sinteticamente ribadire, a nome del Ministro, la disponibilità, anzi la volontà di ricercare e chiedere un confronto, in Aula o in Commissione, quando avremo ottenuto queste definitive conclusioni, sia dell'ENAC che della Commissione di garanzia, per affrontare in un dibattito più compiuto, con elementi probanti abbastanza concreti e oggettivi su cui discutere, l'intera questione, che riguarda non solo i comportamenti dell'Alitalia, ma tutto ciò che concerne gli ostacoli frapposti a questo diritto (che, come dicevo prima, è costituzionalmente garantito) ad una corretta mobilità e ad una corretta informazione sulla mobilità da parte del cittadino viaggiatore e, nel caso specifico, dei viaggiatori che utilizzano il mezzo aereo.

si cerca di sostenere che i disservizi presenti nei trasporti sono unicamente colpa e causa dei lavoratori, che vogliono mantenere assoluti e assurdi privilegi, e delle organizzazioni sindacali che difendono i lavoratori, e non sono per nulla colpa del fatto che in cinquant'anni di storia della nostra Repubblica si è fatto in modo che il senatore Cutrufo citava i pendolari che impiegano due o tre ore per arrivare - l'unico incentivo fosse dato al trasporto privato a scapito di tutto il trasporto pubblico

far sì che la sicurezza dei voli, la ricerca esasperata della competitività, non passasse esclusivamente rispetto a due componenti: in primo luogo la diminuzione dei lavoratori, oltre che la riduzione

facile spiegare che è stato cancellato un volo all'ultimo minuto perché un componente dell'equipaggio all'ultimo minuto si è dato malato. Vorrei chiedere al senatore Cutrufo se sa quanti voli vengono cancellati, e non solo da Alitalia ma dalle dalle compagnie che viaggiano nei nostri aeroporti, per il semplice fatto che non c'è un numero sufficiente di passeggeri; oppure se sa quanti voli vengono cancellati perché Alitalia, sempre in un'ottica di ricerca della riduzione dei costi, ha di fatto dismesso una politica di manutenzione dei propri aerei.

Certo, si può dire che allora era tutta pubblica e che non si badava ai costi; sta però di fatto che Alitalia era additata a livello mondiale come una delle compagnie più sicure, cosa che oggi non è.

e mi pare ci sia stato un impegno che qui ci ha illustrato il Sottosegretario - se una serie di disservizi

non c'è bisogno di invocare la Commissione di garanzia. Il diritto di sciopero nei servizi, soprattutto nel settore dei trasporti, è praticamente un diritto di sciopero virtuale perché tra le franchigie

attraverso diversi piani di ristrutturazione che, di volta in volta, il nuovo amministratore delegato (che veniva individuato come persona dotata di grandi virtù taumaturgiche,

che i costi relativi al personale siano diminuiti, che gli orari di lavoro (quindi i carichi di lavoro) siano aumentati e che la precarietà, anche all'interno della compagnia di bandiera, sia alta. Semmai il problema dei disservizi è un po' altro rispetto a questa cosa: è il fatto che i piani

da questo consiglio di amministrazione con l'unico scopo di realizzare l'alleanza e di vendere la parte in vendita ad Air France, la quale non può tollerare

Se invece, utilizzando la crisi dei trasporti e i disservizi, si vuole sostenere che c'è bisogno di un'ulteriore stretta sul diritto di sciopero all'interno del settore dei servizi, lo si dica chiaramente:

Voglio ricordare che è vero che gran parte del personale è dipendente su Roma; ma per il personale di volo (sia i piloti che gli assistenti di cabina) che opera su che opera su Malpensa il trasferimento da Roma a Malpensa è a proprio carico, non a carico dell'orario di lavoro. Spesse volte gli equipaggi non arrivano e saltano le coincidenze proprio per questa motivazione,

peraltro che, se i regolamenti sono scritti e sono severi (in quanto riguardano la sicurezza dei passeggeri), vadano comunque rispettati.

Debbo però dire che, dalla lettura della mozione-interpellanza, mi pare di poter individuare una certa confusione; sarà forse per mia responsabilità, in quanto non vedo bene le cose. L'estensore della mozione confonde vari piani di problematiche che si intrecciano sulla questione del trasporto aereo. Si parla di scioperi, di scioperi bianchi, di efficienza dei vettori, di efficienza di Alitalia, di organizzazione degli aeroporti, di norme che regolano il trasporto aereo, del codice della navigazione aerea, del problema di Alitalia e della sua crisi più recente, della questione di Malpensa: tutto questo, per così dire, minestrone di questioni diverse

si è interessata al problema di questi abbandoni di attività di una parte del personale, ha rilevato che queste azioni non erano accettabili ed ha anche assunto delle misure nei confronti del personale.

È anche inutile imputare ad Alitalia le responsabilità degli aeroporti: gli aeroporti funzionano bene o meno bene, sono i vettori che transitano negli aeroporti ad avere delle difficoltà.

così come gli altri: il trasporto aereo è una cosa delicatissima, basta poco per metterlo in crisi. Il senatore Cutrufo, che viaggia, sa che anche nel resto del mondo

Azzardo a dire che ciò deriva anche un po' dalle norme, ma noi viviamo sulla base delle disposizioni approvate dal precedente Governo: l'ultimo codice della navigazione è stato modificato nella fase del Governo di centro-destra

le norme che presiedono al sistema del trasporto aereo: mi pare che, insomma, qualcosa si potrà fare. Certo, deve essere chiaro che trattandosi di un sistema ipercomplesso

il sistema del trasporto aereo collassa ovunque, in Italia e all'estero. Quindi la concordia è fondamentale. Tutte le iniziative che si devono intraprendere per risolvere il gravissimo problema di Alitalia devono essere assunte discutendo con i lavoratori, altrimenti si fa peggio,

la situazione della crisi dell'Alitalia, è un punto su cui varrebbe la pena discutere più a lungo. Non è colpa dei lavoratori o degli scioperi la crisi dell'Alitalia. viene da lontano ormai avvitata su se stessa. Siamo stati e siamo vicini ad una condizione di crisi irreversibile e i lavoratori ne sono ben consapevoli. Siamo stati a un passo dal portare i libri in tribunale

sono state riprese le fila del confronto e, sia pure tra alcune tensioni, inevitabili in questa situazione di difficoltà, mi sembra che si cominci ad intravedere qualche punto di intesa

che, per trovare *partner* che intervengano dentro Alitalia, investendo denaro per un piano di sviluppo, è necessario presentare un piano di risanamento dell'azienda, per fare in modo che questo vettore sia appetibile per l'acquirente.

andrebbe contestato in radice, perché comporta una riduzione della presenza di Alitalia nell'aeroporto di Malpensa. Ebbene, a meno di non voler pensare che coloro che dirigono l'Alitalia non capiscono assolutamente niente,

se Malpensa fosse realmente un aeroporto capace di attrarre traffico, non si dovrebbe avere paura se una compagnia come l'Alitalia,

importanti compagnie che verranno a cogliere questo fiore del nostro sistema aeroportuale!

è che gli aerei dell'Alitalia che partono da Malpensa, per poter avere un carico di passeggeri sufficiente a pagare il costo di quel trasporto,

Imporre ad Alitalia di servire Malpensa perché politicamente utile è un ritorno al passato e mi meraviglia che tale questione sia portata avanti da forze politiche che dovrebbero invece operare sul terreno della liberalizzazione del trasporto

Il problema dello sciopero bianco si è trasformato in un dibattito sulla vicenda Malpensa.

Il fallimento della gara su Alitalia ne è la dimostrazione più evidente, ma tale fallimento va considerato alla stregua di un fallimento della politica di Tommaso Padoa-Schioppa,

Questa vicenda dimostra l'assoluta incapacità del Governo di affrontare una questione così delicata. Il rappresentante del Governo ha fornito poc'anzi risposte

C'è l'esigenza di garantire il diritto di sciopero, ma anche quella di garantire i diritti degli utenti che non possono essere sacrificati sull'altare del conflitto sociale nel settore Ciò che non è tollerabile è precostituire una situazione di incertezza che prolunga l'agonia di un'azienda, operando poi quel salvataggio che sarà determinato e operato attraverso l'intervento della solita banca amica.

il Gruppo di Rifondazione Comunista‑Sinistra Europea esprimerà voto contrario sulla mozione presentata dal senatore Cutrufo ed altri, poiché riteniamo che in questa mozione al centro della discussione non ci sia la più ampia problematica che la questione Alitalia pone in termini di rilancio dell'azienda e di piano industriale (peraltro, su questo punto l'8ª Commissione ha già programmato un incontro con l'amministratore delegato dell'Alitalia): dell'Alitalia): in questa mozione si punta esclusivamente il dito sui lavoratori, mentre è ormai evidente che le cause della crisi dell'Alitalia sono da ricercarsi altrove e segnatamente in scelte gestionali e politiche sbagliate. Come se le proteste dei lavoratori siano la causa e non la conseguenza della drammatica situazione che l'azienda sta vivendo. Ci sembra davvero singolare che si condannino i lavoratori, i quali, come si afferma nella stessa mozione, applicano alla lettera norme e regolamenti. Sarebbe necessario chiedersi piuttosto per quali motivi tali regolamenti non vengano normalmente applicati e rispettati in un settore così delicato per quanto riguarda la sicurezza quale quello del trasporto aereo. aereo. Noi riteniamo che se l'Alitalia è giunta a questo punto è perché è mancata in primo luogo la volontà politica di rilanciarla; è mancato un piano industriale serio, che ridisegnasse rotte e flotta, al fine di offrire al cosiddetto sistema Paese uno strumento utile in un settore così delicato quale quello del trasporto aereo. Di questa devastata situazione che viviamo oggi portano la responsabilità i Governi che si sono finora succeduti e le politiche di privatizzazione che gli stessi hanno sostenuto. Le elargizioni generose e gli ammanchi, non sempre giustificati, gli smembramenti, i tagli irrazionali hanno disarticolato l'azienda e hanno finito per indebolire l'Alitalia e per ridurre la sua capacità di stare sul mercato. Non sono mancati i tentativi di svenderla al miglior offerente e al minimo costo. Sotto questo profilo, secondo noi il piano proposto dal consiglio di amministrazione dell'Alitalia reca con sé forse la fine delle speranze di mantenere alla compagnia di bandiera un ruolo significativo. Ciò che il piano propone rappresenta, di fatto, la trasformazione dell'azienda in una compagnia «regionale», con un raggio d'azione limitato, e inevitabilmente destinata a portare acqua ad un altro grande vettore (che sia Air France o Lutfhansa ha poca importanza). Gli effetti sull'occupazione e sul Paese non saranno certo positivi. L'ultima occasione per un vero rilancio, pur con tutte le difficoltà del caso, si è presentata un anno fa, quando il Governo poteva, accanto a un'inevitabile seppur parziale privatizzazione, prospettare un piano industriale, ma ancora una volta la strada scelta è stata quella di un'impostazione meramente finanziaria. E ancora una volta la politica non ha avuto il coraggio di scommettere sul futuro, su un futuro diverso. In definitiva, riteniamo che questa mozione testimoni l'incapacità e l'indisponibilità di una parte della politica - che non ha saputo negli anni trovare risposte adeguate per contrastare la gestione fallimentare di quest'azienda

esigenze legittime e che si trovano a dover pagare drammaticamente una situazione di cui non hanno responsabilità. Noi auspichiamo che l'attuale Governo, in accordo con le indicazioni provenienti dal Parlamento e con lo stesso programma dell'Unione, abbandoni l'approccio e l'impostazione meramente finanziaria a vantaggio di un significativo rilancio dell'azienda, che tenga in massima considerazione la tutela dei diritti dei lavoratori e di conseguenza tuteli anche i cittadini.

che nel dibattito che ne è scaturito si è parlato poco degli scioperi bianchi, o quantomeno si è parlato di coesione sociale,

non siamo però solidali con gli errori del Governo, non siamo certamente d'accordo quando il senatore Paolo Brutti parla delle norme che il precedente Governo

nel senso che si tratta di norme internazionali e non certo inventate dal Governo Berlusconi. Le norme che il Governo Berlusconi ha portato avanti non erano altro che un adeguamento di modernizzazione del sistema, adattando le nostre norme antiquate a norme internazionali.

comandato dai sindacati, con una connivenza politica dove si è privilegiata l'assunzione, si sono abbastanza discutibili sui *catering*, sugli *handling*, su situazioni che hanno portato l'Alitalia, e in linea generale il sistema del trasporto aereo del nostro Paese, fuori mercato.

invece non abbiamo fatto altro che eufemisticamente ricapitalizzare. Coloro che sono veramente professionali sanno però che quando ci sono perdite di un milione - e oggi forse di un milione e mezzo - euro al giorno non si tratta di una ricapitalizzazione: è solamente un continuo fondo perduto per coprire inefficienze, incapacità, mancanza di concorrenza, e quindi

nessun competitore serio internazionale comprerà l'Alitalia con 22.000 persone. Nessuno parla dei reali esuberi; si parla di concordia sociale. Ho sentito anche dire che ogni programma deve essere concordato con i lavoratori.

però in più di un intervento da parte di alcuni colleghi ho sentito affermazioni che ritengo assolutamente inaccettabili. Per parlare bisogna avere conoscenza del problema.

per un volere politico dell'Alitalia, ma certamente non per un volere politico al servizio del nostro Paese. Ho sentito anche

Orbene, da Milano partono 66 aerei con rotta Milano‑Parigi per portare il traffico intercontinentale su Parigi. Questo è un dato che pochi conoscono.

di grandi vettori internazionali che sono disposti a prendere i 150 *slot* che Alitalia ha improvvidamente dichiarato di voler tagliare. Non da ultimo, si è deciso che di 17 voli intercontinentali 14 passeranno da Malpensa

puntiamo su un falso problema, così mi pare abbia detto testualmente il collega Cantoni.

Ha fatto bene il Governo: c'è un fatto preciso? Il Governo si è dimostrato disponibile; anzi, ha cominciato ad attivarsi prima della sollecitazione che è venuta dalla mozione per verificare

veniamo da esperienze nelle quali lo sciopero si fa a viso aperto, guardando negli occhi, cercando di far pagare un prezzo più basso possibile agli utenti e ai cittadini

una forte critica politica ed etica nei confronti di forme di sciopero che non sono accettabili e che colpiscono così duramente i cittadini. Tuttavia il punto è un altro: l'avete posto anche voi intervenendo, non parlando della vostra mozione

efficienza e di continuità del servizio se non affrontiamo i problemi di fondo del trasporto aereo nel nostro Paese? Penso che sia un'illusione. Inviterei i colleghi di Forza Italia, che hanno portato con il loro Governo e i loro alleati la compagnia di bandiera del nostro Paese ad un stato disastroso, a fermarsi lì, prendere atto di questo e vedere come si possa uscire da tale situazione.

prima a Malpensa, poi a Fiumicino (a Malpensa negli anni scorsi, a Fiumicino quest'anno), frutto di un'organizzazione sbagliata in quegli aeroporti e non di norme europee? Trovo molto importante, ad esempio, che il Governo - e non sono solo dichiarazioni, ma vi è un atto formale

che, sulla base di una richiesta del Gruppo dell'Ulivo e delle forze della maggioranza, vogliamo affrontare una discussione concreta e non generica - come in parte è stato fatto - su un altro punto: la riorganizzazione di Alitalia. Per questa ragione, proprio la prossima settimana, su nostra richiesta, è prevista l'audizione dell'amministratore delegato di Alitalia presso l'8a Commissione del Senato. se vogliamo dare una risposta vera ed efficace ai cittadini, di questi punti dobbiamo parlare, li dobbiamo affrontare con un'azione concreta di Governo. Sinceramente la vostra mozione sposta del tutto il terreno e non risponde alla domanda che i cittadini e gli stessi lavoratori di Alitalia ci fanno. Mi dispiace, perché sarebbe stata necessaria, e speriamo sia possibile un'azione convergente per risolvere davvero i problemi veri che abbiamo di fronte.

Pur condividendo le preoccupazioni - come ho già detto in premessa - espresse nella mozione e riaffermando la volontà del Governo, del Ministro di riferire nelle sedi opportune, in Aula o in Commissione, sull'istruttoria posta in essere,

prima di illustrare questa mozione credo sia il caso di fare una brevissima storia del tema in essa perché ci dà il quadro per comprendere anche come taluni fenomeni si sviluppano in agenzie completamente controllate dal Ministero del tesoro, ma che di fatto pongono la politica e il Ministero stesso al margine. Stiamo parlando qui di un concorso del mese di novembre 2005, bandito dall'Agenzia delle entrate, per l'assunzione di 1.500 funzionari. Le prime assunzioni sono avvenute il 22 giugno 2006, data dalla quale è poi entrata in vigore la relativa graduatoria di merito. È importante evidenziare quanto la finanziaria abbia detto in riferimento al mantenimento in vita delle graduatorie di merito, tant'è vero che ha prorogato il termine di scadenza di queste graduatorie fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 1 della citata legge finanziaria, al comma 530, dispone che una parte delle nuove assunzioni di personale dell'amministrazione economico-finanziaria sia destinata alle agenzie fiscali, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione tributaria, richiamando all'uopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, che prevede espressamente «la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate».

dal presidente Benvenuto ai colleghi Bonadonna, Russo Spena, Barbolini, Pegorer, Eufemi, Costa, Curto ed altri, che di fatto denunciavano tale comportamento dell'Agenzia delle entrate.

sia di maggioranza che di opposizione, ad iniziare dal Presidente della stessa Commissione, si è ritenuto soddisfatto), ma l'aspetto più grave è che il sottosegretario Lettieri non ha espresso un parere del Governo sul tema esposto, che richiamava tra l'altro atti e provvedimenti, ad iniziare dalla finanziaria 2007, a leggere un appunto che la stessa Agenzia delle entrate ha fornito al Governo, addirittura ipotizzando che è molto meno costoso indire un nuovo concorso che non attingere ad una graduatoria comunque già attiva (perché i tempi la rendevano attiva), nonostante la stessa volontà politica del Governo

il sottosegretario Lettieri non riusciva a darci notizia che due giorni dopo l'Agenzia delle entrate avrebbe bandito, come ha fatto, un nuovo concorso; di fatto si è creato un *vulnus* vero e proprio. Noi abbiamo evidenziato e sottolineato (mi permetto di dire «noi» perché mi sono buoni testimoni i colleghi che hanno partecipato a quella seduta)

assorbiti ed entrare negli organici dell'Agenzia delle entrate o comunque di altri enti che operano nello stesso settore, per dare una risposta concreta alle aspettative di queste persone,

Signor Presidente, sarò molto breve perché gli argomenti sono sostanzialmente coincidenti con quelli illustrati dal collega Tofani per senatori sullo stesso tema. Peraltro, come è facile verificare, entrambe le mozioni raccolgono firme della maggioranza e dell'opposizione,

le riflessioni contenute nelle due mozioni, possa portare all'approvazione unanime da parte del Senato di un ordine del giorno impegnativo per il Governo. Da questo punto di vista ciò che ci dirà il Governo

sono state risposte alle interrogazioni cui faceva riferimento il senatore Tofani, ed erano insoddisfacenti; c'è stata un'ulteriore interrogazione mia e della collega De Petris al Governo, riferita al fatto che il Governo ci diceva che stava procedendo ad un nuovo concorso all'Agenzia delle entrate e che vi erano difficoltà per formulare una norma che consentisse di chiamare

risultasse vero che, bypassando in qualche modo le norme che prevedono il concorso pubblico per le Agenzie di cui trattassi, si fossero determinate delle assunzioni. In effetti emerse, anche se in maniera molto reticente, che Equitalia - che, essendo una società per azioni, ancorché controllata, non ha l'obbligo dell'assunzione attraverso il concorso - aveva proceduto a soddisfare alcune esigenze di organico attraverso la chiamata diretta, realizzata con una selezione operata da aziende specializzate, attraverso i cosiddetti cacciatori di teste. Dopodiché, ovviamente, abbiamo in qualche modo verificato che questo tipo di assunzione finiva per essere oggettivamente in contraddizione con la disponibilità di personale selezionato e qualificato che era nella graduatoria nella graduatoria degli idonei. Peraltro, mentre si stava discutendo il decreto sull'IVA, noi eravamo giunti ad un'ipotesi di emendamento concordato con il Governo che prevedeva la possibilità di assumere

presentato. Oggi noi chiediamo che, anche in vista della manovra finanziaria, ci sia un impegno serio un impegno serio che consenta di mettere a disposizione di un'operazione necessaria, quale quella del completamento degli

e anche di altre amministrazioni, la possibilità di selezionare e chiamare da questa graduatoria degli idonei, fatta salva ovviamente la congruenza delle specifiche qualità professionali. Non mi dilungo ulteriormente nell'indicare e specificare gli elementi della mozione. Mi pare sia importante a questo punto sapere qual è la posizione del Governo in modo da poter ragionare sul documento conclusivo, sugli atti che il Senato dovrà deliberare.

indicazioni che dal Ministero giungono, si risponde quindi congiuntamente alle mozioni dei senatori Tofani ed altri e dei senatori Bonadonna ed altri in quanto involgono una problematica di analogo contenuto concernente le graduatorie del concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle entrate per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1.500 funzionari per la terza area funzionale - fascia retributiva F1 - per attività amministrativo-tributaria. Con la mozione dei senatori Tofani ed altri si evidenzia in particolare che l'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha prorogato il termine di scadenza delle graduatorie del concorso in argomento al 31 dicembre 2008. L'articolo 1, comma 530, della citata legge finanziaria, nel disporre la destinazione alle Agenzie fiscali di una parte del nuovo personale da assumere nell'ambito dell'amministrazione economico-finanziaria destinato a potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, richiama il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248, che prevede espressamente la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate.

l'articolo 1 della legge finanziaria citata, al comma 544, ha disposto l'immissione in servizio di 300 idonei del concorso per Ispettori del lavoro; Con la mozione dei senatori Bonadonna ed altri viene segnalato che l'Agenzia delle entrate ha indetto una nuova procedura selettiva per l'assunzione di 500 funzionari con contratto di formazione e lavoro, nonostante sussistesse la possibilità di fare fronte all'avvertita esigenza di ulteriori risorse umane mediante utilizzazione delle graduatorie del concorso precedente, indetto in data 25 ottobre 2005, per l'assunzione di 1.500 funzionari, prorogate

Le signorie loro onorevoli chiedono in particolare l'impegno del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati all'assunzione degli idonei in precedenti selezioni sia per l'Agenzia delle entrate sia per le altre amministrazioni pubbliche, tra le quali le Agenzie fiscali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al riguardo, in via preliminare, si osserva che la problematica relativa allo scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico citato negli atti in esame, indetto dall'Agenzia delle entrate per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di 1.500 funzionari per la terza area professionale, fascia retributiva F1, per attività amministrativo‑tributaria, è stata ampiamente trattata nel corso dello svolgimento di documenti documenti di sindacato ispettivo sia presso la VI Commissione della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 4 aprile 2007 (interrogazioni a risposta

presso l'Aula della Camera dei deputati, nella seduta del 18 aprile 2007 (interrogazione con risposta immediata 3-00821), e, da ultimo, presso la 6a Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 18 luglio 2007 (interrogazione a risposta orale 3-00806). L'Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti osservazioni di competenza, aggiornate alla luce dei risultati della prova scritta del nuovo concorso per l'assunzione di 500 funzionari per attività amministrativo-tributaria. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto per l'Agenzia delle entrate un apposito stanziamento per assumere, mediante concorsi, 1.500 funzionari nel 2006 ed altri 500 nel 2007; tali assunzioni sono finalizzate al potenziamento dell'attività di controllo. La prima *tranche* di 1.500 funzionari è stata reclutata a giugno del 2006 al termine di un concorso che prevedeva, per i vincitori, la stipula di un contratto di formazione e lavoro di due anni. Una volta concluso tale periodo, i vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato, se la valutazione del servizio prestato sarà positiva. Un certo numero di candidati risultati idonei in quel concorso hanno chiesto all'Agenzia di non bandire un nuovo concorso per la copertura di altri 500 posti, ma di procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso. A sostegno di tale richiesta, gli interessati hanno addotto ragioni di tipo giuridico e di tipo economico-organizzativo. Dal punto di vista giuridico, essi hanno richiamato l'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che la dotazione di personale delle Agenzie fiscali possa essere potenziata secondo le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 203 del 2005. Al riguardo gli interessati hanno segnalato che, con l'indizione di un nuovo concorso, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto alla situazione dei candidati idonei al concorso per ispettori del lavoro, per i quali il comma 544 della stessa legge finanziaria ha disposto l'immissione in servizio. Sul versante economico-organizzativo, la tesi sostenuta è che lo scorrimento delle graduatorie eviterebbe i costi di una nuova procedura concorsuale, consentendo di coprire subito i posti da assegnare. Per le ragioni di seguito esposte, l'Agenzia delle entrate non ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di scorrimento delle graduatorie e ha bandito il 6 aprile scorso un nuovo concorso per le assunzioni di personale da effettuare nel 2007. La prova scritta si è svolta il 13 luglio. In merito alle motivazioni relative alla scelta di bandire un nuovo concorso l'Agenzia delle entrate ha osservato quanto segue. Sotto il profilo normativo, il concorso per i nuovi 500 funzionari è stato bandito dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 2, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 203 del 2005. Tale disposizione fa riferimento alla possibilità per l'Agenzia di assumere a tempo indeterminato, in deroga al blocco delle assunzioni, personale precedentemente reclutato anche mediante procedure selettive flessibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. È proprio in virtù di tale norma che i contratti di formazione e lavoro stipulati nel 2004 e nel 2005 dall'Agenzia sono stati trasformati lo scorso anno in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Occorre in generale ricordare come l'assunzione degli idonei rappresenti una determinazione discrezionale correlata alla posizione di mera aspettativa allo scorrimento della graduatoria ricorrente in capo al soggetto risultato idoneo in graduatoria. Conformemente alla giurisprudenza costante del giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 settembre 2006, n. 5320, e Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 gennaio 2007, infatti, la regola ordinaria per l'accesso al pubblico impiego è quella di risultare vincitori in un concorso, mentre lo scorrimento delle graduatorie concorsuali costituisce una facoltà eccezionale, espressione di ampio potere discrezionale. Nel caso di specie vi sono precise ragioni di opportunità, di equità, di convenienza costi-benefìci e di potenziamento organizzativo che indicano come la decisione di bandire un nuovo concorso configuri un esercizio corretto del potere discrezionale rimesso all'amministrazione. Occorre precisare che comunque già in una precedente occasione l'Agenzia ha utilizzato le graduatorie degli idonei. Infatti, nel concorso a 744 funzionari (con contratto di formazione e lavoro) bandito alla fine del marzo 2004, i vincitori sono stati assunti a novembre dello stesso anno e subito dopo, a dicembre, sono stati assunti 321 idonei. Anche nel concorso a 950 funzionari svoltosi l'anno precedente la selezione effettuata aveva consentito di coprire solo poco più della metà dei posti a concorso (430 posti sono rimasti scoperti). Sono quindi stati chiamati a copertura dei posti residui 321 idonei, tra i quali gli ultimi 40 sono stati destinati al Dipartimento per le politiche fiscali (che aveva formulato una richiesta in tal senso). La loro immissione si è resa necessaria per coprire almeno una parte del fabbisogno programmato che il precedente concorso a 950 funzionari non aveva potuto soddisfare. Né era ipotizzabile in quel momento (dopo i tagli apportati alla dotazione finanziaria dell'Agenzia) bandire un nuovo concorso, che è stato invece possibile avviare solo un anno (a ottobre del 2005), grazie all'apposito finanziamento previsto al riguardo dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, già citato. L'Agenzia delle entrate ha precisato, altresì, che esistono ragioni di opportunità (migliore selezione), considerato che con l'indizione di un nuovo concorso si è potuto attingere a una platea assai più ampia di potenziali candidati. Nel nuovo concorso che l'Agenzia ha bandito, oltre alle prescritte forme di pubblicità legale, legale, sono state per la prima volta adottate in modo sistematico procedure di comunicazione diretta dell'avvio della procedura concorsuale ai neolaureati delle Regioni interessate con un *curriculum* particolarmente qualificato, in modo da incentivarne quanto più possibile la partecipazione. L'Agenzia delle entrate ha evidenziato, infine, che il giudice ordinario, adito da alcuni idonei per ottenere lo scorrimento delle precedenti graduatorie, ha di recente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, demandando la competenza in materia al giudice amministrativo, che - come sopra riferito - per costante orientamento giurisprudenziale ritiene che le pubbliche amministrazioni, qualora intendano procedere all'assunzione di personale, non sono obbligate a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, ma - nell'esercizio del proprio potere discrezionale - possono decidere di bandire un nuovo concorso. presentata dal senatore Bonadonna e da altri senatori, viene evidenziata inoltre la possibilità che le altre pubbliche amministrazioni attingano alle graduatorie degli idonei di concorsi già espletati dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si osserva quanto segue. Riguardo la possibilità di ricorrere all'applicazione della disposizione normativa, di cui alla citata legge n. 3 del 2003, l'Agenzia del territorio ha rilevato che, per le proprie esigenze di personale, ha già proficuamente attinto alle selezioni effettuate dall'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita convenzione stipulata con quest'ultima, sottoscrivendo alcuni contratti di formazione e lavoro per personale appartenente a specifiche professionalità. L'Agenzia del territorio ha altresì precisato che, tenuto conto del prevalente profilo tecnico e delle carenze localizzate negli uffici del Nord Italia, ove dovessero manifestarsi esigenze di personale nell'area giuridico-amministrativa, l'Agenzia non mancherà di avvalersi delle graduatorie in argomento, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2008, in virtù del citato articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In proposito, l'Agenzia delle dogane ha osservato di aver espresso il proprio parere favorevole in merito all'emendamento 2.0.117,

E il Governo infatti sta rispondendo.

In proposito, l'Agenzia delle dogane ha osservato di aver espresso il proprio parere favorevole in merito all'emendamento 2.0.117, proposto all'Atto Senato n.

nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, a stipulare contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo particolarmente qualificato, da determinare ai sensi di quanto previsto nel secondo periodo del del citato comma 530, nelle graduatorie formate a seguito di procedure bandite dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relativamente alla problematica in esame, l'Agenzia del demanio ha evidenziato che, successivamente alla trasformazione dell'Agenzia medesima in ente pubblico economico ad opera del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, non trovano più applicazione le norme proprie del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. In particolare, l'Agenzia del demanio ha osservato che, a decorrere dal 1° ottobre 2004, data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'Agenzia del demanio-ente pubblico economico, la stessa provvede ad effettuare tutte le assunzioni di personale nel rispetto delle norme nel rispetto delle norme di diritto privato. In conclusione, si deve rilevare come le scelte dell'amministrazione non siano affatto estranee ad una piena considerazione degli interessi legittimi vantati dagli idonei nell'ambito di procedure concorsuali già espletate, interessi da valutare e coordinare con le scelte discrezionali dell'amministrazione stessa. L'avvenuto avvio ed espletamento parziale della procedura concorsuale indetta dall'Agenzia delle entrate non esclude l'opportunità di una valutazione circa eventuali e concrete soluzioni, anche normative, in ordine al futuro inserimento dei soggetti risultati idonei

L'ordine del giorno si pone la finalità di impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa utile anche con l'inserimento nel disegno di legge finanziaria per il 2008 di disposizioni con adeguate risorse finanziarie finalizzate a prevedere l'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici già espletati, per dotare le Agenzie fiscali degli organici necessari a potenziarne le attività antielusive e antievasive e a provvedere affinché altre amministrazioni pubbliche del comparto finanziario,

Presidente, mi limiterò semplicemente ad annunciare il voto favorevole di Sinistra Democratica al dispositivo che è stato concordato e e all'ordine del giorno accolto dal Governo, che abbiamo firmato. Ci sembra infatti che possa essere un avvio di soluzione ad una situazione che si era creata in rapporto alle legittime aspettative

un rapporto di fiducia tra cittadini, amministrazione ed istituzioni, che per tanti aspetti, e soprattutto per l'eccesso di discrezionalità, a volte viene fortemente compromesso. Ribadisco pertanto,

un "compitino" elaborato dal Ministero dell'economia con degli strafalcioni di carattere giuridico che non abbiamo potuto non evidenziare. Non si può affermare in Parlamento che le Agenzie fiscali o delle dogane hanno dato parere su un emendamento.

rispetto al ruolo delle Agenzie, che rivendicano un'autonomia che non possono avere, perché esiste una responsabilità politica del Ministro dell'economia,

ossia una scelta del Parlamento rispetto alla vicenda dei soggetti idonei, è stata portata avanti, anche come affermato dal Sottosegretario, attraverso una serie di giustificazioni che non hanno fondamento,

Abbiamo votato una legge finanziaria e non è stata rispettata la norma in essa contenuta, applicata soltanto per il Ministero del lavoro. L'Agenzia delle entrate si è sottratta alla necessità di affrontare il problema della lotta all'evasione e dell'elusione fiscale attraverso la maggiore dotazione di risorse umane e soprattutto anche tecnologiche. Ciò è indispensabile se vogliamo affrontare la lotta all'evasione in maniera seria. Possiamo infatti vedere che la Regione Lombardia è quella più scoperta rispetto alla dotazione umana, alle risorse umane necessarie. Tale questione va affrontata in maniera corretta, attraverso lo scorrimento delle graduatorie e non con un nuovo concorso che pone una serie di problemi come quelli che abbiamo riscontrato, con ricorsi ai tribunali amministrativi. Noi portiamo tutte le vicende del Paese all'interno dei tribunali. Dobbiamo rivendicare il ruolo della politica e delle scelte di carattere parlamentare, se vogliamo recuperare e non vogliamo scivolare verso questa deriva, che i grilli parlanti portano avanti in maniera certamente poco confacente ad uno Stato democratico. Per quanto riguarda la vicenda su cui abbiamo richiamato l'attenzione, la Regione Lombardia, che è la più produttiva del Paese, quella che ha maggiori entrate fiscali e necessità di personale, non ha questo personale perché si è voluto fare un altro concorso. Lei non conosce la vicenda, Sottosegretario; noi abbiamo già sollevato il problema delle dogane: c'è un'insufficienza di personale nelle aree di maggiore criticità, quali Genova, Napoli, laddove invece abbiamo visto che il personale è stato dirottato in posti dove non è necessario, come per esempio all'Aquila, a Potenza o a Matera per ragioni clientelari. Questa è la situazione del Paese. Allora, come possiamo affrontare il discorso del del contrasto alle importazioni clandestine dalla Cina se non si rafforza la presenza del personale a Napoli, che è il maggiore porto per quanto riguarda quelle importazioni,

A mio avviso, nell'ordine del giorno che stiamo per approvare sarebbe stato necessario un atto di censura verso il direttore dell'Agenzia delle entrate, perché dovrebbe valutare attentamente le conseguenze anche rispetto al danno erariale che si viene a determinare per la pubblica amministrazione attraverso l'indizione di un nuovo concorso, rispetto alla possibilità di contenere i costi attraverso l'assunzione degli idonei,

riteniamo che questa decisione parlamentare che stiamo per assumere possa portare ad un atto di resipiscenza da parte del responsabile dell'Agenzia, che non può mettersi in contrasto contro la volontà del Parlamento. Parlamento. Riteniamo altresì che sia necessario adeguare le risorse finanziarie, come ho sottolineato al senatore Bonadonna, con un ulteriore ampliamento degli stanziamenti, che occorra salvaguardare il diritto all'assunzione degli idonei, in particolare per coloro che si trovano in prossimità del 32° anno, perché un ulteriore differimento delle assunzioni pregiudicherebbe definitivamente, ingiustamente e irreparabilmente la loro posizione.

concretamente il fenomeno. Infatti solo una lotta all'evasione portata avanti in modo serio e attraverso adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria può determinare le condizioni per una riduzione del carico fiscale

in qualche modo, dialogando positivamente con il Parlamento, in questo caso con il Senato, riassume pienamente la propria funzione pienamente la propria funzione e rispetto alle Agenzie, agli organi tecnici, per quanto importanti, impegnativi e sofisticati, si colloca nella posizione giusta dell'organo che governa il Paese, che risponde del suo operato agli elettori e che non oppone ragionamenti di ordine tecnico e tecnicistico non soltanto alle aspettative legittime di giovani che hanno partecipato ad un concorso ma anche ad una domanda più complessa e più complessiva della pubblica amministrazione la quale, peraltro, deve rispondere efficacemente ad un *input* che lo stesso Governo e la stessa maggioranza pone, quello di recuperare l'evasione fiscale. Da questo punto di vista non accetterei in nessun modo un confronto tra l'Aula ed il presidente o il direttore dell'Agenzia delle entrate o di altre Agenzie perché l'interlocutore

rispetto ad una deriva tecnica, tecnologica, tecnocratica che troppo spesso, anziché aiutare chi governa, finisce con il determinare impacci e, soprattutto,

Signor Presidente, nell'ascoltare le dichiarazioni del Governo ci si convince sempre di più di come la società italiana, oltre che complessa, è anche complicata ad una scarsa capacità di governo complessiva fa riscontro una inusuale adattabilità del corpo sociale che riesce ad esprimere una certa vitalità, anche laddove - *horribilis dictu* - rende virtuosa l'evasione fiscale che, comunque, ha favorito la crescita delle piccole imprese, evidente riscontro di una buona parte di responsabilità della struttura burocratica nei confronti dell'evasione fiscale, virtuosa o meno che sia. Ed oggi dalle reiterate dichiarazioni di chi ci governa si vuole mettere freno al fenomeno facendo leva su di una amministrazione fiscale che faccia conto dell'elevata professionalità dei propri componenti i quali possono disporre, fra l'altro, di una massiccia utilizzazione degli strumenti informatici. Auguriamo che ciò possa avere successo; ma conosciamo le origini del problema di metodo sulla «mitologia» della separazione fra ruolo politico e responsabilità amministrativa sorta agli albori della unificazione del nostro Paese e diffidiamo di chi oggi pensa che tale separazione possa essere stata attuata con la creazione delle Agenzie ed in particolare con quella delle entrate, al punto di aver creato una perfetta autonomia di quest'ultima dal potere politico. Ricordiamo che nel periodo liberale della nostra storia politica l'osmosi fra politica e burocrazia divenne naturale come logica conseguenza della circolarità degli incarichi fra funzioni di Governo e funzioni amministrative e il fenomeno produsse una gracilità nelle classi dirigenti al punto che proprio i giuristi liberali acclararono la separazione fra attività amministrativa e direzione politica dell'amministrazione. Separazione che ha superato la sottomissione del periodo del ventennio e ha continuato a fungere da modello anche nel periodo repubblicano che con la vigente Costituzione ha ribaltato il principio della legge n. 100 del 1926, restituendo al Parlamento, con la riserva contenuta nell'articolo 97 della Costituzione, una competenza della quale era stato escluso. Non vogliamo fare la storia della nostra pubblica amministrazione, ma intendiamo riaffermare il nostro ossequio alla Costituzione sul principio della primazia del Parlamento. Dopo aver ascoltato in audizione presso la 6a Commissione finanze e tesoro il Direttore generale delle entrate, pur apprezzando nel merito la funzione svolta contro l'evasione fiscale in continuo con quella esercitata dal passato Governo, non possiamo essere d'accordo circa la sua autonomia sullo svolgimento di un concorso per l'assunzione di 500 nuovi impiegati, quando il Parlamento attraverso atti di sindacato ispettivo ha espresso una unanime volontà di utilizzare per quella esigenza, gli idonei del precedente concorso del 2005. I ruoli debbono essere distinti fra attività amministrativa e direzione politica dell'amministrazione così come è sancito dalla Costituzione. Consentire altro significa tradire l'insegnamento della storia e i principi costituzionali.

e quello doganale è un comparto di estrema delicatezza che comprende non solo la competitività mercantile, ma anche la sicurezza nella sua accezione più generale per il nostro Paese. se ci sono ancora idonei disponibili di quel concorso, poterli utilizzare oltre che per le entrate, anche per le dogane e non certo come soggetti residuali.

il percorso di trasformazione e crescita qualitativa dell'Agenzia delle entrate nell'arco del decennio 1997-2007, tra i materiali che furono distribuiti nell'occasione ce n'era uno che riportava in premessa una citazione da Georges Bernanos: una citazione da Georges Bernanos: «La speranza è un rischio da correre». Ne è evidente e anche appropriato il significato con riferimento all'indubbia positiva evoluzione conosciuta dagli strumenti del sistema fiscale nel nostro Paese in questo decennio e particolarmente per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate: un percorso che torna a merito di chi vi si è cimentato, su cui all'inizio forse non tutti avrebbero scommesso e che oggi ci consente di poterci giovare dei risultati raggiunti. Ma voglio interpretare quella citazione, ovviamente forzandone il senso, anche come riferibile alla questione di cui oggi è chiamata ad occuparsi l'Aula del Senato. Dico questo perché, pur dando atto e riconoscendo una sfera di autonomia con conseguente assunzione delle relative e piene responsabilità alle scelte della direzione dell'Agenzia delle entrate, non mi convincono le argomentazioni di merito che hanno portato la stessa Agenzia a privilegiare l'opzione di indire un nuovo concorso per 500 assunzioni, che saranno disponibili una volta espletate le procedure in corso di esecuzione alla fine del 2007 anziché fare ricorso, in tutto o in parte, alle possibilità di scorrimento della graduatoria relativa al progetto di selezione Iride, graduatoria che la finanziaria ha determinato di mantenere vigente fino alla scadenza del 31 dicembre 2008. Voglio chiarire che non sono insensibile alle argomentazioni che mettono in evidenza la necessità di avere cura di non discriminare i laureati nel frattempo affacciatisi sul mercato del lavoro rispetto alla data di svolgimento di quel precedente concorso. Né considero fuori luogo la preoccupazione di trovare le migliori condizioni, atte a garantire il rafforzamento degli organici in modo duraturo, nelle sedi del Nord Italia, dove maggiori sono i volumi di attività, gettito e necessità di accertamento. Ma queste esigenze non sarebbero state contraddette da un ricorso allo scorrimento della graduatoria cui ci si riferisce. Se non erro, infatti - cito ancora fonti dell'Agenzia delle entrate - solo in una prospettiva di mero mantenimento della capacità operativa attuale vi è la necessità per l'Agenzia, oltre che la previsione, di rimpiazzare le oltre 3.100 unità in uscita nel prossimo triennio con almeno altre 1.600 assunzioni, oltre le 500 già deliberate per questo 2007. E tutti noi sappiamo, e come Gruppo dell'Ulivo condividiamo, che occorre operare un investimento ulteriore in termini di risorse umane qualificate se vogliamo rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Anzi, è proprio a questo riguardo che mi sembra debole la giustificazione che si sarebbe agito da parte dell'Agenzia in forza di ragioni di opportunità, di equità e di convenienza costi-benefici perché mi pare, invece, si sia rinunciato ad impiegare risorse che sarebbero state immediatamente operative ed utilizzabili già nel corso del 2007 e che si sarebbe potuto costruire una migliore pianificazione dei tempi e della tempistica per acquisire anche ulteriori competenze e figure professionali con un processo, quindi, che avrebbe dovuto graduare e valorizzare l'insieme delle assunzioni e delle risorse umane, senza mortificare - lo dico chiaramente - aspettative di giovani che giustamente non sanno spiegarsi il perché di atteggiamenti contraddittori dello stesso Governo che per alcune sfere di attività ha fatto la scelta di utilizzare le graduatorie di idonei esistenti e per altri ambiti, come in questo caso, ha deciso finora di avvalersi di nuove procedure, lasciando inascoltate quelle aspettative e quelle richieste. Ma torno, per concludere, signor Presidente, al punto da cui sono partito: la speranza è quella di aprire con la discussione di questa sera una prospettiva di soluzione e la scelta è quella di correre il rischio - permettetemi di dire così - di poter verificare di qui a qualche tempo di aver potuto avere, sulla base di questa prospettiva, anche l'esito efficace di un risultato concreto. Lo sottolineo: come Gruppo dell'Ulivo vogliamo sperare che la discussione di oggi ed il voto all'ordine del giorno che ci accingiamo a dare contribuiscano a costruire quella prospettiva positiva per trovare una soluzione. Del resto, il Governo nel percorso di costruzione del disegno di legge n. 1485 e nel lavoro d'interlocuzione con la nostra Commissione, aveva lavorato con noi, nella persona del sottosegretario Grandi, cui va dato atto di quell'impegno, ad una norma di sblocco della situazione, prevedendo anche la possibilità che altre amministrazioni e Agenzie (penso ai problemi delle dogane che sono stati richiamati e del territorio o altri settori nella sfera della pubblica amministrazione finanziaria) potessero attingere a quelle graduatorie. Non se ne fece niente anche per problemi di copertura finanziaria, oltre che per l'esito di quel provvedimento. Ma l'intenzione c'era e positiva, e oggi l'ho ritrovata. Ho fatto un po' fatica nel percorso di lunga ricostruzione, ma nella parte conclusiva dell'intervento del rappresentante del Governo ho ritrovato quella determinazione e quella disponibilità sulla base, quindi, di un'apertura circa un impegno nella direzione che avevamo auspicato e prefigurato. Poiché siamo nell'imminenza della presentazione della finanziaria e la lotta all'evasione fiscale è una priorità del Governo, oltre che un'emergenza nazionale e tutto il sistema delle Agenzie è carente di personale qualificato per compensare il *turn over* e allinearsi alla complessità degli adempimenti richiesti dalla situazione sempre più pressante, ci sono tutte le condizioni per andare nella direzione concreta che abbiamo cercato di determinare, partecipando e contribuendo a questa discussione. Voteremo come Gruppo dell'Ulivo a favore dell'ordine del giorno, con la speranza - ma, voglio dirlo al rappresentante del Governo, anche con la tenacia - che si determini una prospettiva risolutiva del problema.

intervengo per dichiarare il dissenso dal mio Gruppo e per annunciare un voto di astensione in quanto ritengo che l'approvazione di tale ordine del giorno costituisca una soluzione molto più sfumata rispetto a quella della mozione presentata dal senatore Tofani e

se non di spontanea volontà con atti di indirizzo predisposti dal Ministero, avrebbe dovuto ottemperare a quanto disposto dalla legge finanziaria. Non facendo ciò viene meno, non solo per insipienza ma secondo me con comportamenti che rasentano